ai magistrati che sono stati oggetto dello spionaggio denunciato dal Consiglio superiore della magistratura, quella mia personale e dei senatori del Gruppo della Sinistra Democratica.

secondo la quale egli avrebbe detto: «Io ho una cultura industriale e per me il CSM è il Centro sperimentale metallurgico, che è anche una cosa più seria». La frase è virgolettata. Siccome non posso credere che il portavoce unico del Governo l'abbia pronunciata, segnalo in questa sede l'opportunità di una smentita. aggiungere che la Commissione giustizia ha appena deliberato di richiedere al CSM l'invio della delibera assunta a questo riguardo, in modo che il Parlamento possa assumere le eventuali iniziative consequenziali. del giorno - ma non ne siamo molto distanti - un Ministro di questo Governo, che si occupa per la verità (o perlomeno dovrebbe occuparsi, in base alla tabella che ho letto degli incarichi ministeriali) di materia diversa dalla giustizia,

Ricordo a questo Ministro che il lavoro parlamentare, corretto anche se serrato e contrapposto, l'esame e la votazione degli emendamenti non rappresentano un inciucio, ma il sale della democrazia, di quella cultura democratica della quale forse qualche esponente del nostro Governo non è pienamente dotato. Vorrei aggiungere, altresì, che nessun attacco all'indipendenza della magistratura è contenuto nell'eccellente disegno di legge che abbiamo al nostro esame, tant'è vero che lo stesso Ministro in questione, in una lettera resa nota alla stampa inviata al ministro Mastella, chiede di intervenire su tre punti, commettendo su due di questi uno strafalcione. Si potrebbe dire «e che ci azzecca?», volendo usare una terminologia di questo tipo. Nella prima chiede di modificare una norma che era stata già modificata nel senso da lui posto; nella seconda chiede di modificarne un'altra che è stata stralciata (forse bisognerebbe spiegare a questo Ministro che lo stralcio vuol dire che si esamina il testo in una fase successiva); nella terza chiede di modificare - in questo starebbe l'attacco all'indipendenza della magistratura - una disposizione, per quanto riguarda la distinzione delle funzioni, in modo che, invece che lo spostamento da corte di appello a corte di appello, lo spostamento avvenga da Regione a Regione. È una questione che riguarda pochissime Regioni italiane. È difficile vedervi un attacco all'indipendenza della magistratura, anche perché - come ha fatto notare il senatore D'Ambrosio - nessuno costringe un magistrato a cambiare funzione; per citare le sue parole: «Se non vogliono cambiare distretto, evitino di mutare funzione». Mi permetterà, signor Presidente, onorevoli colleghi, di dare più peso ai consigli e alle indicazioni del senatore D'Ambrosio che a quelle del Ministro in questione. Per il disegno di legge che stiamo esaminando, in effetti, ci si propone (ed anche per questo abbiamo giustamente operato), rispettando ovviamente la posizione contraria espressa in più occasioni rese ancora ieri con il voto sulla pregiudiziale dell'opposizione, in un clima che non sia di scontro frontale, perché noi vogliamo che ci sia un ordinamento giudiziario che resti nel Paese, che non sia modificato ad ogni nuova legislatura, e soprattutto abbiamo cercato di operare al fine di realizzare un ordinamento giudiziario non costruito dal punto di vista della magistratura né da quello dell'avvocatura (ancorché si tratti di interlocutori importanti), piuttosto dal punto di vista del cittadino, che è il trascurato in questo dibattito: abbiamo cercato di costruire un ordinamento giudiziario in cui sia tutelato il cittadino. prevede che ci sia la separazione delle carriere (che al di là di ogni considerazione di merito sarebbe impossibile, come la senatrice Rame sicuramente sa, a Costituzione invariata), ma una distinzione delle funzioni in quanto è interesse del cittadino avere davanti a sé un giudice il giudice il più possibile imparziale e che appaia tale. È una conseguenza di una norma di grande civiltà introdotta nella Costituzione italiana e presente nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella Carta dell'Unione Europea: il principio del giusto processo. Il cittadino ha diritto a che sia distinta la funzione di chi indaga dalla funzione di chi giudica - non si tratta di una richiesta o di una pretesa del potere politico, ma di un diritto che ha il cittadino - naturalmente, nel più rigoroso rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza di entrambe le funzioni. Vorrei che qualcuno si alzasse, qui, dire quale norma sull'ordinamento giudiziario, nel testo mirabilmente illustrato dal relatore Di Lello, possa apparire compressiva dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Così come è diritto del cittadino avere dinanzi a sé un magistrato professionalmente preparato: questa riforma dell'ordinamento giudiziario segna un passo importante in questa direzione per due norme significative che abbiamo introdotto, quella sulla quale mi esprimerò brevemente, di esposizione, inerente al concorso di accesso, che è un concorso di secondo grado, in quanto si richiede una fase preliminare di ulteriore preparazione professionale, e l'altra, fortemente e giustamente voluta dal senatore D'Ambrosio, per la quale nessun magistrato può svolgere funzione monocratica se non dopo aver operato quattro anni in un'attività di collegio ed aver avuto una valutazione professionale a questo riguardo. Perché ancora una volta è il cittadino ad avere diritto che il magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, sia professionalmente preparato e abbia acquisito quel minimo di esperienza professionale anche sul campo, che gli consenta di evitare il più possibile,

è una scelta che mi sento di condividere fino in fondo. Naturalmente, come tutte le leggi, può essere migliorata in questa occasione, potrà essere migliorata successivamente, ma su punti, su ritocchi, su aspetti, non sull'impianto che è estremamente persuasivo. Vorrei aggiungere ancora che, per quanto riguarda la dibattuta questione del ruolo dell'avvocatura, la Commissione ha effettuato una scelta, a mio avviso condivisibile, anche se c'erano colleghi che avrebbero preferito, secondo l'antico programma della sinistra e di Magistratura democratica, la presenza diretta degli avvocati nei Consigli giudiziari: si è ritenuto preferibile seguire una soluzione diversa, che però - attenzione - non è quella di eliminare il ruolo dell'avvocatura, ma di prevedere la procedimentalizzazione del parere che viene espresso dal Consiglio dell'Ordine. Questo vuol dire che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati in sede autonoma - quindi, non partecipando al confronto diretto con la magistratura - fornirà, ai fini delle valutazioni che i Consigli giudiziari devono dare e trasmettere al Consiglio superiore della magistratura, un suo parere, del quale il Consiglio giudiziario non potrà non tener conto, se non altro perché se non ne tenesse conto il provvedimento assunto sarebbe suscettibile di difetto di motivazione e quindi impugnabile in diverse sedi. sedi. Questa scelta, quindi, consente all'avvocatura (non dal punto di vista dell'interesse di una corporazione, ma dal punto di vista di una categoria di professionisti che, oltre a svolgere la loro attività professionale, esercitano anche la funzione estremamente importante di garantire il diritto dei cittadini alla difesa, previsto

che questa attività di esercizio del diritto alla difesa trova intralci in comportamenti poco professionali o poco preparati della magistratura, di fornire un suo rapporto del quale il Consiglio giudiziario dovrà tener conto ai fini della valutazione dell'attività dei magistrati. Tutto ciò non è per nulla compressivo dell'autonomia di alcunché. Ricordo che richieste di questo tipo furono a suo tempo formulate dalla stessa magistratura associata, alla quale naturalmente va la nostra stima e il nostro sostegno

di magistrati in attività non propriamente legali; ecco se forse, esaurita la doverosa attenzione alla riforma dell'ordinamento giudiziario, l'Associazione nazionale magistrati si occupasse anche di questi fenomeni, darebbe un contributo all'attività che tutti noi in Parlamento vogliamo svolgere per un miglior funzionamento della giustizia italiana e dell'ordinamento giudiziario. Questa non è una legge contro nessuno, è il tentativo di fare una legge dal punto di vista del cittadino, quindi cercando di capovolgere la logica fin qui seguita da parte di tutti, chi più, chi meno, di affrontare il tema della magistratura come se si trattasse di un conflitto tra magistratura e sistema politico o di un conflitto tra magistratura ed avvocatura. Abbiamo provato a fare una legge

ripeto, perfettibile e migliorabile come tutte le cose umane - questa legge possa restare salda. E ci auguriamo che anche quella che oggi è l'opposizione - che dal suo punto di vista legittimamente si oppone, voterà contro, e così via - voglia tener conto che stiamo dando una base nella quale riteniamo che la parte non strumentale, la parte non legata a interessi di Tizio o di Caio, che sappiamo benissimo essere presenti, raccolga una giusta questione di garantismo (che non è una bandiera della destra, perché storicamente il garantismo è stato una bandiera della sinistra, ma deve essere comune a tutto il Parlamento). Con questa riforma dell'ordinamento giudiziario abbiamo ritenuto delle preoccupazioni che vengono da quella parte, nella misura in cui da ciò non derivasse - come in alcun modo deriva - la compressione di quei fondamentali princìpi di autonomia ed indipendenza della magistratura che costituiscono un pilastro immodificabile della democrazia italiana come voluta dal Costituente.

Signor Presidente, si è da più parti affacciata la preoccupazione di un accordo strisciante, che sarebbe in atto tra maggioranza e opposizione - e di cui francamente continua a sfuggirmi "il movente" - teso a consentire un'indolore trasformazione in legge del disegno di legge con cui il Governo e la maggioranza di centro-sinistra hanno in animo di impedire che la riforma dell'ordinamento giudiziario, studiata e democraticamente votata nella passata legislatura dalla maggioranza di centro-destra, diventi - a sessant'anni di distanza dalla relativa prescrizione costituzionale - definitiva "cosa fatta". Premesso che non posso far altro che rassicurare chiunque ne dubiti sul fatto che nessuna pulsione autolesionistica ha improvvisamente attraversato alcuno di noi, di noi senatori della Casa delle Libertà, né che alcuna utilità di giornata ha determinato alcun cambiamento di rotta rispetto alla nostra volontà di modernizzazione del nostro sistema giudiziario, anticamera vera e necessaria, anzi indispensabile, per restituire quell'efficienza di sistema che oggi manca e che è, ad ogni occasione, oggetto di una declamazione inutile e ormai anche un po' stantia sui ritardi nelle procedure, sui buchi di riservatezza e quant'altro, e quant'altro, sfiderò il pericolo di essere anch'io sospettato di "trama" o di "accordo sottobanco" con la maggioranza, ma non intendo sottrarmi al dovere di riconoscere, e non per semplice motivo forma, la qualità del lavoro svolto dal senatore Di Lello Finuoli e l'onestà intellettuale da lui tenuta nel suo ruolo di relatore nelle diverse fasi attraverso cui il detto lavoro si è snodato nel corso di queste ultime settimane in Commissione giustizia. Dico questo per anche subito aggiungere che primo e inescusabile torto di questo Governo e di questa maggioranza risiede nella non accettabile ristrettezza dei tempi imposti per trattare una serie di materie peraltro e per giunta inizialmente proposte nelle forme, vere e proprie, del provvedimento *omnibus*. Il Senato avrà, infatti, avuto a disposizione, al termine del dibattito, poco più di tre mesi per discutere la materia dell'ordinamento giudiziario, la materia dell'accesso in magistratura, delle carriere dei magistrati, delle loro - nuovamente virtuali - valutazioni, della scuola della magistratura e di quant'altro. Alla Camera dei deputati resteranno invece una decina di giorni, se vorrà rispettarsi il termine stabilito dalla legge, che Governo e maggioranza - e non altri - hanno inteso a suo tempo presuntuosamente individuare nella data del 31 luglio 2007. A meno che già non sia A meno che già non sia nella riserva mentale di essi, l'idea di ricorrere al Capo dello Stato, perché questi si costringa a misurarsi con il monito, ancora poche settimane fa fermamente ribadito dalla Corte costituzionale, sottoscrivendo un decreto-legge di proroga che sarà palesemente privo di qualsiasi contenuto di impellente necessità e urgenza, così come prescritto dall'articolo 77 della nostra Costituzione, posto che nessuna vacanza di legge vi sarà, se il provvedimento oggi in esame non fosse approvato entro il detto termine della fine del mese, alla luce del fatto che il decreto legislativo attuativo della riforma Castelli, che delle stesse questioni si occupa, potrà in quel caso nuovamente spiegare i suoi effetti. Quattro mesi in totale, dunque, per esaminare, discutere e dibattere quanto, nella passata legislatura, è stato oggetto di centinaia di riunioni, di migliaia di ore di studio e di impegno, nell'arco continuativo di quasi quattro anni, giudicati - e "urlati" - dall'allora opposizione di centro-sinistra e dai vertici dell'Associazione dei magistrati come "un tempo senz'altro esiguo e insufficiente". Credo al riguardo di poter dire che "senza vergogna" è l'unico corretto modo per qualificare la condotta, di allora e di oggi, dell'una e degli altri, e che quindi - proprio per questo - torna la necessità di svolgere un ringraziamento al relatore per quanto e per come egli ha fatto, così da consentire - questo è stato il risultato del suo impegno - una quanto meno accettabile soglia di dignità e di qualità del nostro lavoro. Proporrò ora alcune riflessioni generali sul provvedimento, riservandomi di completare le stesse, illustrando di volta in volta gli emendamenti presentati e dichiarando il relativo voto. La prima riguarda la questione della separazione delle carriere, quella - e non solo - per cui gli avvocati - vedendosene allontanare l'attuazione - in questi giorni scioperano, astenendosi dalle udienze.

di dover cambiare casa d'abitazione, a causa dell'obbligo di trasferimento fuori della regione di residenza, così come è stato previsto in sede di Commissione giustizia. La mia personale convinzione è da sempre stata quella della necessità di intervenire in tal senso, per un'effettiva separazione delle carriere fra i giudici e i magistrati del pubblico ministero, conseguenza ed evoluzione ordinamentale naturale dopo la riforma costituzionale del "giusto processo", del giudice terzo e imparziale, ma - fermo ciò - ho anche sempre trovato indubbia la necessità del percorso costituzionale per pervenirvi. Ne sono persuaso ora, ed ero di ciò persuaso anche nella passata XIV legislatura, quando di questo si parlò in termini maggiormente concreti rispetto al passato, e quando non esitai a sostenere la tesi, a fronte dell'allora contingente impraticabilità di una riforma costituzionale per la mancanza delle relative condizioni politiche, dell'obbligo di attestarsi su una rigorosa separazione delle funzioni. Così come poi è stato e come è nella previsione contenuta nella cosiddetta riforma Castelli. Il programma con cui il centro-sinistra si è presentato al Governo del Paese dopo le elezioni del 2006, so bene che non ha mai previsto - né avrebbe mai potuto pretendere di prevedere alcuna ipotesi di separazione delle carriere tra giudicanti e requirenti, né - tantomeno - progetti di armonizzazione del sistema del pubblico ministero secondo conformi modalità, come stabilite in altri Paesi europei, né per quanto riguarda la questione del controllo della polizia giudiziaria, né per quanto riguarda la questione - anch'essa collegata - dell'obbligatorietà (in realtà, signor Presidente, della discrezionalità) dell'azione penale nel nostro Paese. Paese. Del complesso di tutte queste questioni, infatti, occorre congiuntamente dibattere, e non indistintamente di ciascuna di esse, con la necessità di soluzioni globali, che tengano conto di tutti gli aspetti in ragione della loro complementarietà e della necessità della oculata apposizione di opportuni pesi e contrappesi. La separazione delle carriere dei magistrati non era dunque attesa, ma nemmeno ci saremmo mai potuti attendere un ritorno al passato della misura cui ora assistiamo: perché qualche temperamento vi è stato rispetto alla prospettazione iniziale di puro e semplice ripristino del previgente sistema incentrato sulla totale e duratura promiscuità, ma non granché. granché. Si potrà forse andare un po' in là, se saranno approvate nostre proposte di ulteriore modifica, ma se sarà invece approvato l'emendamento del senatore Brutti si potrà tornare anche più in qua. Non dovrà infatti più cambiare Regione il magistrato che vuole cambiare funzione se, essendo requirente, accetterà di svolgere mansioni civili: disfatta organizzativa annunciata per i tribunali di minori dimensioni e per chi ancora sostiene che non debba esservi disparità di trattamento tra nessuno. Ma si tratta di un argomento che non appassiona, perché anche in questo caso l'uniformità di trattamento corrisponderebbe al diritto di un singolo giudice, mentre l'inverso sarebbe smacco per la collettività dei giudici in politica che, della promiscuità delle funzioni, hanno fatto uno slogan conclamato e, a parere mio, un totem indifendibile nel tempo. la valutazione delle carriere, vi è odore di piena restaurazione, quindi, come del resto è per un'altra centrale questione, quella della progressione in carriera dei magistrati e del connesso procedimento di valutazione. Nessuna pretesa che quanto scritto nella cosiddetta riforma Castelli fosse esente da difetti o da imperfezioni. Anzi, secondo accreditate correnti di pensiero, troppo timida fu quella riforma e, aggiungo anche, poco sostenuta dalla stampa l'azione riformatrice della Casa delle libertà e, conseguentemente, poco apprezzata dalla stessa opinione pubblica che, correttamente informata, non avrebbe esitato - ne sono convinto - ad approvare il superamento di leggi come legge Breganze o Breganzone. Leggi che hanno affermato per i giudici (e solo per i giudici, un vero *unicum* nel Paese) il principio dei "*todos caballeros*", azzerando ogni riferimento a merito, a capacità, a laboriosità. Nessuna pretesa di perfezione della riforma Castelli, dunque, nella parte cui ora mi riferisco, e forse, addirittura, la necessità di correzione ancora prima che la stessa fosse in concreto sperimentata. Ma mai ci saremmo attesi una restaurazione violenta come, malgrado qualche temperamento postumo, sarà quella che uscirà dal testo in esame. I giudici, ancora una volta solo i singoli giudici, saranno nuovamente indifesi ostaggi dei loro colleghi più potenti, secondo uno schema che è diventato collaudatissimo nel tempo. I giudici, ancora una volta, solo i singoli giudici, appiattiti sulle volontà altrui (altro che indipendenza ed autonomia), anche se, per la verità, non obbligatoriamente: basta infatti che rinuncino alla più banale aspirazione, che è quella di fare un po' di carriera o di avere un incarico di prestigio o semplicemente desiderato e il problema non sarà più sussistente. Molto semplice, insomma: "essere nessuno", in cambio di un po' di libertà. Ciò secondo uno schema che è ben collaudato e che ha il suo centro (ancora mi asterrò dal dire la sua cupola) in un Consiglio superiore della magistratura, che ha dimenticato da tempo la missione costituzionale alta che l'articolo 105 ad esso assegna, per trasformarsi in una banale proiezione pantografica delle correnti dell'Associazione nazionale magistrati: iattura vera del sistema, perché lungi dal rappresentare una virtuosa occasione di pluralismo, ne costituisce solo palestra del compromesso politico. Compromesso politico ancor più basso nel rango, allorché sono da proteggere interessi altolocati, o - piuttosto - da assicurare impunità quando vi è travalicazione dei compiti

il magistrato che (quantomeno - va riconosciuto - senza il demerito dell'ipocrisia e della banalità) aveva impartito istruzioni all'ufficio da lui diretto di contravvenire ad una legge testé varata dal Parlamento, in una materia così delicata, come quella dell'indulto e della sicurezza dei cittadini.

Solo così si può infatti spiegare la marcia indietro del Governo e della maggioranza sulla presenza degli avvocati nei consigli giudiziari. In qualsiasi sistema moderno la valutazione di funzionamento di un servizio e di chi lo presta è fornito da chi se ne avvale, cioè dai clienti. Non così è il sistema della giustizia, che evidentemente mal sopporta le parrucche, quando si tratta di dirlo, ma certamente non quando si tratta di farlo. E così non dovranno valutare proprio nulla i clienti, cioè i cittadini o, meglio, i loro rappresentanti naturali, che sono nel nostro caso gli avvocati, dapprima chiamati ai consigli giudiziari, primi luoghi di valutazione, e poi espulsi con motivazioni balbettanti, perché né vere, né sentite. Infatti, le motivazioni vere e sentite della timorosa retromarcia della maggioranza sono in realtà quelle, ancora una volta non dicibili, rappresentate dal pericolo di *vulnus* al "patto della dettatura" tra maggioranza e Associazione nazionale magistrati (dopo quello "della crostata", in sede politica, quello "della macchina da scrivere" in sede giudiziaria). Il presidente Salvi ha cercato di dare spiegazioni, cercando di giocare, per così dire, in contropiede; ma egli non ha saputo e non ha potuto spiegare l'infondatezza di quanto all'opposto si è detto circa la non nocività della presenza semplicemente istituzionale dei presidenti dei consigli dell'ordine, che sarebbe stata minore del dovuto. quanto si è detto in ordine ai conflitti tra magistrati ed avvocati, che o non contano nulla oppure sono destinati ad essere patologia e come tali regolati. Nessuno - come si è detto - può smentire la circostanza che dei consigli giudiziari sono parte i pubblici ministeri, che proprio in funzione di quella riforma costituzionale dell'articolo 111 sono parte nel processo e non magistrati a tutto titolo. stralci. Ho prima parlato di un disegno di legge *omnibus*, un vero e proprio assalto alla diligenza da parte degli ambienti più disparati, e con l'affermazione delle pretese più diverse e stravaganti. Delle stesse, i colleghi hanno modo di vedere che è stato fatto ampio strame, attraverso numerose proposte di stralcio che sono avanzate all'Aula. Non voglio trasformare questo mio intervento in un discorso "contro", soprattutto in un discorso contro il Consiglio superiore della magistratura; ma tra i tanti assalti alla diligenza, dei quali già peraltro la Commissione ha reso giustizia, ne va ricordato uno e cioè anche quello, singolarissimo, del Consiglio superiore della magistratura, che, pur di asservire a se la scuola della magistratura (che invece sarà utile, e non carrozzone ulteriore, solo se autonoma e indipendente), si era fatto singolarmente affermare la propria competenza anche in relazione alle attività di formazione dei magistrati stranieri, e all'organizzazione dei sistemi giudiziari di altre nazioni. Come se ad esso - e non al nostro Governo - possa competere la prerogativa di regolare la politica estera (perché anche l'assistenza giudiziaria di altri Stati è politica estera) del nostro Paese. Ma vi è tra le norme di cui è proposto lo stralcio, e di cui io fermamente continuo a chiedere la soppressione, anche una disposizione che, malgrado sapientemente occultata nella cripticità del testo, non dovrebbe mancare di far discutere non tanto per il suo concreto peso (la nostra Italia è sopravvissuta a ben altro), ma perché la dice lunga sulla disinvoltura di taluni. Si tratta del comma 51 dell'articolo 6, mirante ad assicurare ai magistrati dai 40 anni in su, che viaggiano per ragioni di servizio, il diritto di utilizzare in aereo la prima classe. Mi permetto di sorridere pensando all'assordante silenzio giornalistico di chi, anche di recente, si è disinvoltamente (irresponsabilmente?) avventurato nella via della denuncia dei costi della politica, che devono essere inesorabilmente puniti, se sono sperperi o abusi di una politica cialtrona, ma che in realtà corrispondono a costi della democrazia, in ogni altro caso, e dunque assai pericolosi, nel momento in cui si desidera cancellarli, con buona pace di chi si professa «professionista» dell'etica. Ma a parte il sorriso, introduco l'argomento solo perché sono colto da un dubbio, signor Presidente. La disposizione in esame è di quelle che comportano una spesa o no? Gli aerei sono gratis per i magistrati? O paga l'Alitalia? O paga, invece, lo Stato, tanto per cambiare? Non sono mai stato un esperto di bilancio, ma credo di poter dire che la domanda sia retorica. La disposizione citata, ove mai fosse stata approvata, avrebbe certamente comportato una spesa: piccola o grande, poco importa. E mi chiedo, allora come è possibile che, della detta spesa, non si sia avveduta l'attenta Ragioneria che produce le schede tecniche per la spesso bacchettante Commissione bilancio del Senato:

A meno che non vi siano due Ragionerie e due Commissioni bilancio: una Commissione bilancio quando governa l'onorevole Prodi e una per il centro-destra. al ministro Di Pietro, signor Presidente, il Consiglio superiore della magistratura ha ieri, ancora una volta, dato unanime dimostrazione (l'unanimità è, in questo caso, la prova ulteriore di un disvalore) di quanto sia conclamata la sua predisposizione a travalicare le proprie attribuzioni, e in questo caso l'ha fatto (ma non è la prima volta) cercando i riflettori dell'attualità. Il Consiglio superiore della magistratura ha infatti compiuto un esercizio oggi assai di moda, che è quello di processare il nostro servizio segreto militare e il suo precedente vertice. L'ha fatto, peraltro, mostrando a tutti come non si fanno i processi, cioè giungendo ad affermare verità senza ascoltare ogni parte, ogni voce, ma limitandosi ad attenzioni e prospettazioni parziali e conclamatamente di parte. Questo già la dice tutta, con grande malinconia, per chi - come me - aveva affidato grandi speranze di «aria nuova» alla consiliatura in corso. E questo già la dice tutta, anche con buona pace del nostro ex presidente Mancino, che - in veste originalmente minimalista - ci ha spiegato ieri che le risoluzioni non sono sentenze. Di surrealità in banalità. Di banalità in surrealità. Ma tant'è, la cosa è molto piaciuta al ministro Di Pietro che ieri sera, pur sul terreno amico - ma, in questo caso, occorre anche dire intelligente e corretto - di RAI 3, non ha mancato di iscriversi al relativo campionato di surrealità e di banalità nel denunciare anch'egli «le spie» (mah!) e nel difendere i suoi ex colleghi magistrati, presso i quali non so poi di quanta considerazione egli goda. Ma la questione potrebbe poi essere proprio questa. Quel Di Pietro che, a fronte delle proteste (quanto di comodo, non sfugge ad alcuno) dell'Associazione nazionale magistrati, ha subito detto che lui non voterà mai il disegno di legge del nemico-collega Mastella di (non abbastanza) controriforma dell'ordinamento giudiziario e che, tuttavia, mai farà cadere il Governo. Il che vuol dire che voterà la questione di fiducia, se la stessa sarà posta (e ci avrebbe invero sorpreso la sorpresa, nel caso contrario). Non so come andrà a finire, Presidente, e non so se la questione di fiducia sarà effettivamente posta. Non so, per la verità, come andrà a finire e se, una volta posta la stessa per l'ennesima volta, essa ancora sarà registrata nel Senato e in Parlamento; probabilmente sì, ma non certo nel Paese, perché i cittadini la fiducia l'hanno persa da un pezzo e non è certo con provvedimenti di qualità polverosa e stantia, come questo, che se ne potrà recuperare. Neanche un po'.

giudiziario arriva, devo dire, con toni molto smorzati: nel Paese non se ne ha quasi notizia, eppure la voglia e la domanda di giustizia sono elevate.

discussione. Purtroppo in televisione non si vedono più i film di Totò; ma è un altro Totò nazionale che ravviva ogni tanto la scena con qualche battuta o qualche bel siparietto:

di ruolo. Abbiamo persino il nuovo senatore Gerardo D'Ambrosio che critica i colleghi. Passata la barricata,

ma anche lo *status* di intoccabili. Oggi, se qualche politico o qualche giornalista prova a criticare un magistrato,

la sovranità popolare. C'è anche qualche collega che, per avere la paginetta sul giornale, promette tagli e fa proposte di legge di tagli alle pensioni e quant'altro. Poi lo stesso collega che fa queste proposte

qualche minaccia di sciopero non degli avvocati (che giustamente qualche dritto lo avranno anche, in questo Paese) ma da parte dei magistrati e subito la politica ha trovato una veloce corsia preferenziale;

vorreste cancellare la vocina delle vostre promesse elettorali di togliere lo scalone. Ha già cominciato D'Alema a dirlo, ma sono sicuro che, se si potesse fare un *referendum* segreto magari qualcuno della sinistra estrema - tra i banchi della Margherita, passando dai DS e dallo stesso D'Alema, si direbbe che la riforma Maroni voi l'avreste fatta uguale. L'avreste fatta uguale e votata e, se possibile, l'avreste tenuta. Ma per rientrare

di valorizzare l'aspetto sistematico della normativa ed il pericolo della riforma Castelli. Effettivamente, il quadro normativo in materia di ordinamento giudiziario (che la relazione al disegno di legge richiama effettivamente in maniera compiuta) ha subìto diversi interventi disomogenei, d'urgenza, anche pasticciati, che dimostrano la necessità, proprio con la riforma Castelli, di un percorso che porti efficienza, efficacia, elimini la burocrazia, risponda, nei limiti del possibile, alle domande di giustizia dei cittadini e di certezza del diritto di tutti coloro che operano o che ne sono coinvolti, nel mondo forense. Questa riforma, a nostro giudizio, non risponde a queste esigenze; anzi rappresenta la continuazione di quel percorso normativo che la stessa relazione criticava. Nelle parole questa maggioranza illustra un'esigenza, ma poi nei fatti - ed è questo che conta - si comporta in maniera scomposta, incapace di affrontare i problemi.

Non parliamo, signore e signori, di un disegno di legge che stabilisce un principio blando, ma parliamo di una riforma che coinvolge tutti i cittadini e, quindi, della democrazia in questo Paese. è stato questo dibattito, quindi, con la richiesta di un disegno sistematico per creare una disciplina tale da garantire maggiore funzionalità ed efficienza. Mai in passato, però, così tanti segnali critici e di preoccupazione. Abbiamo già citato le dimissioni della giunta esecutiva dell'Associazione nazionale magistrati; l'Unione delle camere penali sciopero "di fronte alla protervia" - addirittura - "di chi vuole conservare l'esistente ed impedire una riforma democratica dell'ordinamento giudiziario e mortifica l'avvocatura". Non mi che sembra sia un segnale di entusiasmo da parte del Paese. Domani saranno i cittadini a protestare per una giustizia burocratizzata, immobile, incapace di dare risposte. Il disegno di legge contiene alcuni passaggi definiti da tutti inaccettabili e peggiorativi: se c'è chi parla di inciucio, noi possiamo dire, invece, che ci troviamo di fronte ad un pasticcio napoletano, vista la Regione di appartenenza del Ministro. Riporto le considerazioni che provengono dal mondo forense per sottolineare il clima di forte critica: "Viene messo in campo un progetto di matrice autoritaria, statalista e illiberale che delinea la magistratura come potere autocratico, autogovernato ed autoreferente, forte ed invasivo, in grado di dettare le regole

magari più sotto la spinta delle intercettazioni che di un'effettiva preoccupazione, parla di un rischio per la politica.

D'Alema. Un disegno di legge, quindi, che nasce, viene modificato, viene influenzato secondo logiche inaccettabili in tema di valori, princìpi costituzionali e certezza del diritto e che dimostra una politica debole, incapace di volontà riformatrice, ma spinta dalla necessità semplice e ben palese ben palese di abbattere la riforma Castelli. Occorre invece, a nostro giudizio, procedere nello spirito della riforma avviata nella scorsa legislatura, che abbatteva il vetusto ordinamento giudiziario Grandi (mi sembra evidente che dopo sessant'anni sia legittimo modernizzare l'assetto legislativo), capace di disciplinare l'assetto della magistratura e reggere il confronto con la realtà degli uffici della giurisdizione.

l'accesso in magistratura ripropone l'unicità dell'accesso mediante concorso ordinario e cancella la verifica di idoneità psico-attitudinale prevista nella riforma Castelli. Non si comprende la *ratio* di tali scelte e soprattutto perché i magistrati, che svolgono una funzione rilevante e delicata, debbano essere esentati dall'idoneità psico-attitudinale. Presidente, nella vita faccio il neuropsichiatra e ho fattotest attitudinali per caldaisti, vigili, persone che chiedono il porto d'armi, personale militare: forse che un caldaista svolge un mestiere più pericoloso e più necessario di equilibrio

con un minimo di test psico-attitudinali sarebbe stato possibile individuare determinate caratteristiche oppure tendenze psicologiche. La paranoia,

Le proposte in tema di valutazione della professionalità contenute nel disegno di legge in discussione si ricollegano, sia pure con alcune novità, alle disposizioni contenute nel disegno di legge presentato dal ministro della giustizia Flick all'epoca del I Governo Prodi. Ma non volevamo dare un segnale di rottura con il passato? Signor Presidente, appare dubbia l'efficacia dell'obbligatorietà della formazione. Il disegno prevede che tutti i magistrati frequentino almeno un corso di formazione ogni quattro anni. Tutti noi sappiamo che un periodo temporale di quattro anni è decisamente lungo e inidoneo a garantire un perfezionamento nelle conoscenze giuridiche (soprattutto quando si limita l'aggiornamento ad un corso solo). Analoghi dubbi nutriamo sul percorso di verifica. Viene previsto un sistema di valutazioni, con verifiche ogni quattro anni, dove la valutazione della professionalità è fatta dal CSM. Oh, mamma mia: il controllore e il controllato, tutti assieme appassionatamente, come al solito! Vi è un'eccessiva burocratizzazione, che coinvolge anche il sistema dell'autogoverno della magistratura, sistema nel quale sono ormai strutturalmente inseriti i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione. Circa il concorso per magistrato ordinario, scompare l'obbligo di indicare la funzione prescelta. Permane la semplice distinzione dei magistrati invisa), a seconda delle funzioni esercitate, con l'abolizione dell'obbligo iniziale di scelta definitiva tra funzioni giudicanti e requirenti. La stessa cosa avviene in altri Paesi, dove - mi sembra - il tasso di democrazia e di rispondenza alle esigenze dei cittadini non viene martoriato fino a questo punto. Non viene così recepita la separazione delle funzioni prevista dalla riforma Castelli, che diventava definitiva dopo cinque anni dall'ingresso in magistratura, dopo l'obbligo iniziale di scelta definitiva tra la funzione giudicante e quella requirente. Siamo tutti consapevoli della necessità di interventi legislativi capaci di assicurare professionalità e funzionalità all'agire dei giudici e dei pubblici ministeri, garantendo la necessaria imparzialità imparzialità e la necessaria autonomia. Occorre prevedere controlli affinché tale autonomia e indipendenza non diventino mai privilegio, garantendo però al tempo stesso la presenza di un giudice terzo ed imparziale. Questo disegno di legge invece, a nostro giudizio, rappresenta un'offesa ai valori costituzionali dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, incrina le garanzie dei cittadini ad ottenere la certezza del diritto, indebolisce il diritto dei cittadini ad essere uguali

un «no» deciso a questa riforma, un «no» motivato e consapevole, un «no» a quello che questo Governo e questa maggioranza di sinistra stanno compiendo.

Poiché non sono presenti in Aula i restanti senatori iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Conseguentemente, la prevista seduta antimeridiana del prossimo martedì 10 luglio non avrà più luogo.

presso le stazioni di Padova e di Mestre. In quella occasione, i cosiddetti disobbedienti del Nord-Est, guidati da Luca Casarini, che intendevano raggiungere Roma per manifestare contro la visita del presidente americano Bush, hanno mandato in *tilt* tutta la circolazione ferroviaria del Veneto e dell'Alta Italia, bloccando le stazioni di Mestre e Padova. Infatti, i manifestanti *no global*, ai quali si erano uniti anche i «no Dal Molin», ossia comitato che si batte contro l'ampliamento della base statunitense di Vicenza, hanno invaso i binari ferroviari e pretendevano di fatto di raggiungere la città di Roma senza pagare un regolare biglietto. A questo punto, il traffico ferroviario di tutto il Veneto è impazzito ed è rimasto paralizzato per circa quattro ore, con migliaia di passeggeri tenuti in ostaggio nelle stazioni. Pendolari e viaggiatori, rimasti in balia di questa masnada di facinorosi, hanno subito gravissimi disagi e ritardi ed hanno cominciato a chiedere, anche attraverso le associazioni dei consumatori, di essere adeguatamente risarciti per i gravi danni subiti.

Trenitalia ha altresì spiegato che queste erano le «identiche condizioni che offriva per ogni altra manifestazione sindacale o politica». Si tratta di 55 biglietti,

Trenitalia ha inoltre dichiarato che i treni che sono poi rientrati dalla stazione Tiburtina - per i quali non è stato pagato alcun biglietto - sono stati messi a disposizione dei manifestanti *no global* manifestanti no global «su formale richiesta del dipartimento pubblica sicurezza del Ministero dell'interno» ed ha precisato che per il viaggio di ritorno dalla stazione Tiburtina «i manifestanti non hanno pagato il biglietto»; Anche questa circostanza, è però rimasta avvolta nel dubbio, in quanto il prefetto Serra, sempre a mezzo stampa, ha smentito che mai ci fosse stata una richiesta in tal senso rivolta dal citato Dipartimento del Ministero dell'interno a Trenitalia. Trenitalia. Le domande che il sottoscritto intende porre al Governo in questa occasione sono le seguenti. Intanto, vorremmo capire quali iniziative, anche di tipo giudiziario, siano state assunte nei confronti di Casarini, dei *no global* e dei "no Dal Molin", che si sono resi responsabili del reato, evidente a tutti gli effetti, di interruzione di pubblico servizio; non capiamo, inoltre, perché questi disobbedienti, questi facinorosi si rendano protagonisti in diverse occasioni di atti illegali e poi non vengano mai perseguiti in modo adeguato. Vogliamo anche sapere perché le forze dell'ordine non siano immediatamente intervenute quando il blocco del traffico ha cominciato a manifestarsi, non abbiano disperso i facinorosi e abbiano così impedito il blocco del traffico. È del tutto evidente che 150-200 persone, se opportunamente contenute e respinte dalle Forze dell'ordine, non sono certamente in grado di bloccare il traffico ferroviario di tutta l'alta Italia.

ai consumatori che ingiustamente, senza colpa, hanno subìto gravi disagi debbano essere sensibili e tangibili. Inoltre, vorremo sapere a quanto ammontano, ad oggi, le richieste di risarcimento avanzate a Trenitalia da parte dei viaggiatori per quale motivo siano stati stampati a Padova e pagati da Trenitalia solo 55 biglietti ferroviari, a fronte di circa 150-200 manifestanti che hanno raggiunto Roma; per quale altra grande manifestazione sindacale o politica Trenitalia abbia stampato solo 55 biglietti alla tariffa di 10-20 euro per la tratta ferroviaria in questione; se i vagoni ferroviari su cui hanno viaggiato i manifestanti siano stati danneggiati; per quale motivo il Dipartimento pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha chiesto a Trenitalia di mettere gratuitamente a disposizione dei manifestanti no global un treno speciale per il viaggio di ritorno dalla stazione Tiburtina. **Interrogazione sul contingente militare

La questione esposta nell'interpellanza del senatore Zanettin è all'attenzione del Governo, come è testimoniato sia dall'ampia informativa resa presso l'Aula della Camera dei deputati dal vice ministro vice ministro dell'interno, onorevole Minniti, nella seduta del 19 giugno scorso, sia dall'intervento del sottosegretario per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, onorevole Naccarato, in risposta all'interpellanza urgente presentata dall'onorevole Cannavò. Pertanto, anche in questa sede, si riferisce quanto è stato reso noto nelle occasioni appena menzionate, sottolineando peraltro che gli aspetti riguardanti le scelte gestionali ed organizzative di Ferrovie dello Stato e quindi di Trenitalia Spa non sono suscettibili di diretto controllo da parte del Ministero dei trasporti, che è titolare delle funzioni di vigilanza sullo svolgimento dei servizi ferroviari. Nel pomeriggio del 9 giugno, a Roma, durante la visita in Italia del Presidente degli Stati Uniti d'America, si sono svolte due manifestazioni pubbliche: una a piazza del Popolo, promossa dalla FIOM-CGIL e da altre associazioni, con la partecipazione di circa 500 persone, ed un'altra promossa dal Comitato 9 giugno. Al fine di predisporre un regolare trasporto dei manifestanti in arrivo a Roma già nelle giornate del 7 e dell'8 giugno, Ferrovie dello Stato Spa ha tenuto apposite riunioni per valutare l'entità dei probabili flussi, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'interno. Ciò ha consentito di predisporre un piano di assistenza alla clientela per limitare possibili disservizi derivanti dall'occupazione di binari da parte dei manifestanti, in particolare per la zona di Bologna, dove era prevista una concentrazione di circa 600-700 persone, oltre ad altri manifestanti provenienti da località confluenti. Il piano di assistenza prevedeva: individuazione delle aree critiche (Triveneto, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania), individuazione dei referenti per le aree di criticità, individuazione dei treni critici; predisposizione di 58 servizi sostitutivi su gomma dislocati nelle città maggiormente interessate dai flussi di traffico dei partecipanti alla manifestazione (Milano, Firenze, Bologna, Torino, Genova, Roma e Napoli); particolare assistenza ai viaggiatori disabili a bordo dei treni coinvolti, nonché l'individuazione delle comitive coinvolte (circa 350 clienti) al fine di suggerire possibili alternative di viaggio ovvero effettuare, in caso di turbative alla circolazione, il trasbordo sui servizi sostitutivi con bus. L'evoluzione dei flussi di traffico dei partecipanti alla manifestazione è stata monitorata dalla società ferroviaria a partire dalle serate di giovedì 7 e venerdì 8. Dalla serata di venerdì 8 giugno sono stati registrati i primi movimenti nell'area di Trieste, mentre dalla Lombardia e dal Piemonte non sono state segnalate particolari criticità per i treni in partenza verso il Sud nella stessa giornata di venerdì. Sin dalle prime ore di sabato 9 giugno, sono stati segnalati i movimenti dei manifestanti da Trento, Rovereto e Verona verso Bologna. I manifestanti erano muniti di biglietti per treni regionali acquistati alle emettitrici *self service*. Poco dopo, altri movimenti sono stati segnalati a Mestre e Padova. La mattina del 9 giugno, nella stazione di Padova, Trenitalia e le Forze dell'ordine hanno effettuato un'azione di "filtro", a seguito della quale sono stati emessi e pagati sottobordo complessivamente 95 titoli di viaggio con destinazione Roma, aggiuntisi ai biglietti già acquistati dalle persone presenti sul treno attraverso i canali di vendita ordinari. Si rappresenta che è possibile quantificare il numero di biglietti emessi in occasioni precedenti solo a fronte dell'indicazione di riferimenti temporali precisi. Trenitalia ha sempre comunque richiesto il pagamento del biglietto in linea con i prezzi previsti e applicati secondo la normativa vigente e questa ferma presa di posizione ha comportato come conseguenza l'occupazione dei binari di Mestre e di Padova con ricadute sulla circolazione ferroviaria nella zona; tuttavia, i viaggiatori interessati dai blocchi sono stati riprotetti mediante l'impiego degli autobus sostitutivi. La situazione si è sbloccata solo quando i manifestanti hanno accettato di pagare i prezzi previsti per comitiva; analoghe operazioni, senza che si fossero verificati blocchi dei binari, sono avvenute nelle stazioni di Firenze, Genova, Bologna, Pisa, Livorno e Ancona. Al termine della manifestazione, circa 300 persone sono giunte presso la stazione ferroviaria di Roma Tiburtina, presidiata da contingenti delle Forze dell'ordine, mostrando l'intenzione di ottenere una riduzione del biglietto per il rientro a Milano. Dopo lunghe trattative con Trenitalia Spa e numerosi atti di protesta da parte dei manifestanti, che hanno reso necessario l'intervento delle forze di polizia, è stato organizzato il deflusso ed il rientro nei luoghi di origine dei partecipanti ai cortei. Infine, alle ore 1,30 circa, i manifestanti sono partiti a bordo dei due treni speciali messi a disposizione da Trenitalia su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza per evidenti e gravi ragioni di ordine pubblico. Nelle stazioni di Roma Termini, Roma Tiburtina e Roma Ostiense sono stati posizionati appositi "filtri", congiuntamente con le Forze dell'ordine, al fine di consentire il passaggio esclusivamente ai manifestanti in possesso del titolo di viaggio. Nella notte tra il 9 e il 10 giugno, mentre erano in corso gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, è pervenuta alla sala operativa delle Ferrovie dello Stato la disposizione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per la ripartenza dei manifestanti. A seguito di tale disposizione è stato, in particolare, approntato un treno straordinario e i manifestanti sono stati quindi accompagnati alla partenza senza esigere il titolo di viaggio. Per quanto è avvenuto presso la stazione Tiburtina, ad opera di consistenti gruppi di persone, Ferrovie dello Stato spa ha precisato che si sono verificate situazioni critiche dopo l'ennesimo fermo rifiuto del personale della società di consentire il viaggio di ritorno senza il regolare pagamento. Invero, le tariffe applicate in questa occasione sono state quelle relative all'offerta "comitive ordinarie", che offre una riduzione del 20 per cento disponibile presso tutte le biglietterie di stazione del territorio nazionale. Il cosiddetto servizio di controlleria a bordo dei treni è stato svolto dagli addetti con le consuete modalità. Ancora una volta, è opportuno ribadire che nessun manifestante è giunto a Roma gratuitamente, nella scrupolosa osservanza di una pratica consolidata e rispettosa della legge e dei regolamenti ferroviari che si ripete in simili occasioni. I disservizi derivanti dagli eventi connessi alla manifestazione del 9 giugno 2007 sono attribuibili a responsabilità esterne all'Impresa ferroviaria e, pertanto, il risarcimento degli eventuali danni conseguenti non può gravare sulla medesima. In relazione, all'evento in questione, secondo le notizie fornite da Ferrovie dello Stato spa per quanto riguarda i reclami, ne risultano pervenuti a Trenitalia, complessivamente, 19 e per alcuni viene avanzata anche la richiesta di rimborso del titolo di viaggio, mentre per ciò che concerne i danni arrecati al materiale rotabile risultano danneggiate alcune carrozze del treno Milano-Roma, con un costo di ripulitura quantificato in circa 2.500 euro.

assolutamente insoddisfatto anche dei contenuti della risposta che mi è stata fornita, che evidentemente ha natura solo formale, ma non tiene conto dei problemi.

che sotto diverse sigle pone in essere atti vandalici ed illegali, puntualmente annotati dalla stampa e in qualche occasione anche dalle interrogazioni parlamentari di chi vi parla, senza che nessuna autorità si prenda mai la briga di porre fine a queste scorribande? I nomi dei protagonisti sono sempre i soliti, li conoscono tutti, tanto che il loro *leader*, Luca Casarini, viene invitato in alcune occasioni negli studi RAI per pronunciare i suoi strampalati proclami. Perché allora le aggressioni continuano, senza che né magistratura, né autorità di pubblica sicurezza agiscano con la necessaria fermezza? Perché a nessuno dei responsabili è mai stata irrogata una sanzione esemplare? Il blocco delle stazioni di Padova e Mestre si sarebbe potuto evitare se solo ci fosse stata una minima azione di repressione da parte della forza pubblica. Al contrario, queste bande di teppisti di fatto possono contare su un tacito consenso delle Autorità preposte; godono di una sostanziale impunità, inaccettabile di fronte alla stragrande maggioranza dei cittadini onesti che rispettano le leggi. Come al solito, due pesi e due misure. Basti pensare alla repressione subita invece qualche giorno fa di fronte a Palazzo Chigi dai pensionati che protestavano contro il Governo. Con i *no global* guanti di velluto, contro i pensionati invece pugno di ferro! Non credo di sbagliare se dico che voi del Governo vi dimostrate forti con i deboli e deboli con i forti. In secondo luogo, questo Governo ha proclamato in varie occasioni di voler perseguire una politica a favore dei consumatori. consumatori. Il ministro Bersani cerca addirittura di accreditarsi di fronte all'opinione pubblica come il paladino delle liberalizzazioni e dei consumatori. Ma allora, onorevole vice ministro De Piccoli, perché il Governo non ha previsto nessun adeguato risarcimento per tutti quei cittadini pendolari e viaggiatori che, transitando per le stazioni di Mestre e Padova, hanno visto i propri programmi sconvolti nella giornata del 9 giugno scorso? Appuntamenti saltati, ansia e stress determinati da ritardi di ore nella partenza dei treni non meritano forse di essere ristorati in modo non simbolico? Signor Vice ministro, la politica a favore dei consumatori non si fa con leggi *spot* o propagandistiche, come il decreto Bersani, che riduce i costi di ricarica dei telefonini, salvo consentire alle compagnie telefoniche corrispondenti aumenti delle tariffe. Una politica a favore dei consumatori non si persegue indirizzando Alitalia, come state facendo, nelle mani di Air One, un *partner* senza risorse né industriali, né finanziarie, creando sul mercato nazionale un monopolio a danno degli utenti del servizio aereo. Pensate piuttosto a riconoscere sostanziosi risarcimenti in caso di interruzione del servizio ferroviario, come nel caso che oggi stiamo discutendo, o di altri pubblici servizi. Lasciate fallire un carrozzone come Alitalia, che da anni brucia risorse pubbliche. Non prendete in giro la gente, non vendete fumo! Punto terzo e concludo, signor Presidente. Facciamo pagare a tutti i biglietti ferroviari. Il ministro Padoa-Schioppa parla molto dell'evasione fiscale, un male che affligge il nostro Paese. Ma la cultura della legalità va perseguita a tutti livelli. Allora diamo il buon esempio, partendo dalle cose più elementari. Quindi, cominciamo col far pagare a tutti il biglietto ferroviario e magari anche quello dell'autobus. Lo Stato non deve accettare soprusi, né da parte dei *no global*, ma neppure dei pendolari napoletani organizzati, che qualche giorno fa hanno paralizzato la stazione Tiburtina a Roma per non pagare il biglietto ferroviario. Basta anche con le tariffe compiacenti per sindacati e gli organizzatori di manifestazioni: più Stato di diritto e meno arbitri anche su questo fronte. Ma credo che queste ragionevoli richieste non potranno che rimanere lettera morta fino a che al Governo ci saranno le frange estreme della sinistra, Caruso compreso. La riprova di ciò sta nel fatto che avevo proposto di sottoscrivere la mia interpellanza anche ad una collega veneta della Margherita, la senatrice Rubinato; ma questa, anche perché così consigliata dai senatori Treu e Giaretta, alla fine ha preferito declinare l'invito. Probabilmente era troppo imbarazzante per lei e per gli altri esponenti del centro-sinistra condividere con noi questi banali ed ovvi principi di convivenza civile.

L'interrogazione in discussione, prendendo spunto da imprecisate "fonti di stampa" che avrebbero affermato che il nostro contingente in Afghanistan

dell'interrogante, per una scelta irresponsabile del Governo i nostri militari si potrebbero venire a trovare con un equipaggiamento inadeguato in caso di attacco nemico, In ordine all'equipaggiamento del contingente italiano, il Governo ha avuto già modo di riferire, in risposta all'interrogazione 3-00496, presso la 4a Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica, in data 11 aprile 2007. 2007. Sulla questione in esame è opportuno precisare che la valutazione-monitorizzazione della minaccia, sia quella relativa ai nostri militari in Afghanistan che quella riguardante altri contesti d'impiego fuori area, è un'attività fondamentale nel processo decisionale attuato dai singoli comandanti di contingente, allo scopo di individuare le linee d'azione più idonee al conseguimento degli obiettivi assegnati. Di conseguenza, ove a giudizio di un comandante in teatro le risorse umane e materiali a sua disposizione si rivelassero inadatte a fronteggiare l'incombere l'incombere di una determinata minaccia, il vertice tecnico-militare della Difesa rappresenta a quello politico la necessità di adottare le dovute contromisure, atte a garantire la sicurezza e l'incolumità del personale militare italiano. Il Governo, riguardo al tema della sicurezza e della protezione del contingente in Afghanistan, ha assunto sempre un atteggiamento di grande responsabilità e piena consapevolezza dei rischi e dei pericoli connessi alla missione in quel Paese. L'Esecutivo non ha mai trascurato l'aspetto relativo alla necessità che il nostro personale impiegato in Afghanistan venisse dotato di equipaggiamenti, mezzi e materiali adeguati a fronteggiare le minacce e i rischi legati al delicato impegno in quel teatro operativo. A questo proposito, infatti, il Governo ha già adottato alcune iniziative per fornire ai nostri militari tutti gli equipaggiamenti aggiuntivi necessari per farli operare al meglio e nella massima sicurezza nello svolgimento dei compiti assegnati. Tali iniziative, come è stato illustrato dal ministro Parisi nell'ambito delle comunicazioni rese alle Commissioni riunite 3a e 4a del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il giorno 15 maggio 2007, sono state recepite anche in ottemperanza a quanto previsto nei diversi ordini del giorno, adottati sia alla Camera che al Senato in occasione del voto sul finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni militari internazionali all'estero. In proposito, è utile ricordare anche l'attività di raccordo svolta dal Consiglio supremo di difesa nel corso della riunione del 2 aprile scorso nell'ambito dell'analisi della situazione relativa ai vari teatri operativi, in vista delle iniziative che il Governo stesso avrebbe dovuto assumere per attuare quanto previsto dai predetti ordini del giorno. A seguito di tale riunione, il Dicastero della difesa ha interessato immediatamente lo Stato maggiore della Difesa per un esame accurato delle scelte e delle richieste tecniche analizzate dagli Stati maggiori, in relazione alle nuove esigenze da soddisfare, nonché dei relativi ulteriori costi. Sulla base di tali esami, è emersa l'esigenza di dotare il nostro contingente di mezzi che potessero ampliare le capacità di muoversi e operare in sicurezza, grazie ad una combinazione di elevata velocità di reazione, elevata mobilità in ogni contesto orografico, elevata protezione, ampia disponibilità di sensori di sorveglianza ed identificazione, anche a grande distanza; incrementare la sicurezza operativa grazie al loro effetto di deterrenza. Sulla base di questi criteri, sono stati individuati i seguenti equipaggiamenti: elicotteri A-129 "Mangusta", di cui uno come riserva logistica; otto veicoli corazzati "Dardo"; dieci veicoli blindati "Lince". Gli elicotteri A-129 sono velivoli agili e ben protetti, dotati di sistemi di osservazione ogni-tempo, che permettono di scortare gli elicotteri da trasporto già presenti in teatro, nonché di esplorare il terreno nel quale operano le nostre pattuglie a terra. I corazzati "Dardo" sono veicoli dotati di una valida combinazione di mobilità e protezione, grazie al moderno complesso motore-trasmissione-cingoli ed alla pesante corazzatura. Vista la virtuale assenza di strade nella Regione di Herat, i "Dardo" danno la possibilità ai nostri militari di muoversi con adeguata protezione anche fuori strada e sui percorsi più impervi. gli ulteriori dieci blindati "Lince", caratterizzati da una specifica protezione antimina, aumentano la sicurezza delle nostre pattuglie in movimento sulle rotabili. Nel recente passato tali mezzi, già presenti in teatro, hanno dimostrato la loro capacità di resistere alle esplosioni di ordigni improvvisati. Insieme ai nuovi mezzi, sono stati inviati in Afghanistan gli equipaggi ed il personale di supporto tecnico e logistico. Le decisioni assunte - va ribadito - in tutta evidenza non alterano in alcun modo né la natura della partecipazione del nostro contingente alla missione ISAF, tanto meno, le finalità ultime della nostra presenza. Ove si abbiano presenti la dimensione geografica della Regione di nostra responsabilità e le sue caratteristiche orografiche, si comprende come gli equipaggiamenti aggiuntivi, per numero e tipologia, non potrebbero consentire un genere di missione differente da quella già adottata dal nostro contingente, in accordo con gli alleati della NATO. I nuovi mezzi permettono, però, di migliorare le capacità di esplorazione, la mobilità e la protezione (quindi, la sicurezza attiva e passiva) delle nostre truppe. Fatta questa necessaria precisazione, per quanto riguarda, invece, la preannunciata «offensiva talebana di primavera», si fa osservare che essa sta coinvolgendo principalmente le aree Sud ed Est del Paese e soltanto marginalmente le forze nazionali schierate a Kabul ed Herat. Risulta, pertanto, che soltanto le forze della coalizione operanti nelle aree Sud ed Est dell'Afghanistan abbiano incrementato le tipologie di armamento a disposizione. Nelle aree della capitale, Nord ed Ovest del Paese, le unità presenti, in virtù di una situazione al momento maggiormente calma e standardizzata, sono configurate principalmente per condurre attività volte alla ricostruzione, per garantire la *force protection* del personale impiegato e reagire contro possibili offese portate da gruppi di elementi ostili. In conclusione, nel ribadire che i mezzi e gli equipaggiamenti aggiuntivi sono già a disposizione dei nostri militari in Afghanistan, si assicura che il Governo continuerà a dare il massimo sostegno,

un *reportage* a firma di Gianluca Di Feo, si denunciava proprio la scarsa dotazione di armamento difensivo posto a disposizione del nostro contingente schierato in Afghanistan, a fronte di una temuta offensiva talebana che si sarebbe sviluppata nei mesi a seguire. La risposta che oggi ci viene fornita - che in parte c'era stata già stata anticipata dalla stampa e da altre fonti in nostro possesso - ci rassicura, nel senso che, a distanza di quattro da quella denuncia, il tempo non è passato invano e, nel frattempo, è stato adeguatamente e significativamente potenziato l'armamento messo a disposizione dei nostri soldati schierati in quel teatro di operazioni. Ringraziando Dio, poi, in questi mesi, nonostante l' aggravarsi degli scontri che hanno interessato la zona Sud dell'Afghanistan, i nostri militari sono riusciti a sfuggire agli attentati che hanno invece mietuto tante vittime tra gli altri contingenti alleati.

che, in occasione del dibattito parlamentare sul rifinanziamento della missione militare in Afghanistan, ha chiesto, con un proprio ordine del giorno, che quella delicata missione potesse essere proseguita nelle migliori condizioni di sicurezza dei nostri soldati, attraverso un adeguamento del dispositivo bellico posto a loro disposizione.

Non possiamo tuttavia nascondere, signor rappresentante del Governo, che forse, però, oggi le maggiori preoccupazioni devono rivolgersi non tanto al contingente in Afghanistan, ma a quello dislocato nel Sud del Libano, sotto la guida del generale Graziano. Siamo tutti rimasti profondamente turbati dall'attentato terroristico che ha colpito i militari spagnoli, che partecipano alla stessa missione, e che ha provocato otto morti e numerosi feriti gravi.

adeguatamente ragguagliato e informato. Ricordo, a tal proposito, che il decreto-legge relativo alla proroga delle missioni militari all'estero, prevedeva che i Ministri degli esteri e della difesa,

Ed il Governo, ahimè, non ha ottemperato, fino ad oggi, a questo proprio dovere e non sappiamo ancora quando ciò potrà avvenire. Io credo che sia assai grave che, in un contesto di crisi internazionale su temi così importanti, il Governo sia inadempiente e manchi ai propri doveri. In questo caso, mi rivolgo anche alla Presidenza, facendo mia una richiesta che è stata formulata anche da altri parlamentari del mio schieramento politico, invitando la Presidenza a farsi parte diligente nei confronti del Governo perché questo dovere, che è istituzionale e giuridico, perché sancito da un decreto-legge convertito in legge, venga adempiuto al più presto. È del tutto scorretto e inaccettabile che il Governo, fino ad oggi, disattenda a questo

a tre giorni dal rapimento di padre Giancarlo Bossi, nel corso di un'informativa urgente alla Camera dei deputati in Aula, avevo assicurato che il Governo avrebbe tenuto costantemente informato il Parlamento sugli sviluppi del rapimento. Ho accettato quindi con piacere e non solo per dovere istituzionale di essere qui questa sera per fornire un quadro aggiornato sugli ultimi sviluppi del caso. Le circostanze di fatto sono conosciute, non mi dilungherò su di esse. Come noto, padre Giancarlo Bossi, del Pontificio istituto missioni estere (PIME), è stato rapito a Zamboanga City, domenica 10 giugno, mentre si recava a celebrare messa in un villaggio vicino. Purtroppo, non si tratta del primo missionario italiano rapito a Mindanao, dato che negli ultimi dieci anni la stessa sorte è toccata a padre Benedetti, rapito nel 1998 per tre mesi (e sottolineo tre mesi) e a

Come ho avuto modo di segnalare a giugno, la zona in cui è stato rapito padre Bossi è considerata da anni ad alto rischio ed è fortemente sconsigliata dalla Farnesina, anche sulla base delle verifiche effettuate *in loco* dall'unità di crisi. I missionari del PIME hanno sempre fatto prevalere lo spirito di servizio su ogni altra considerazione e non hanno mai abbandonato l'area, come ha fatto padre Bossi privilegiando il suo impegno e la sua missione. La Farnesina ha mantenuto fin dai primissimi momenti del sequestro contatti regolari con le autorità dello Stato della Città del Vaticano e direttamente anche con il PIME per assicurare la piena collaborazione e l'assistenza per la soluzione della vicenda. Tanto l'unità di crisi quanto la nostra ambasciata a Manila, che è in contatto con il nunzio apostolico *in loco*, *in loco*, monsignor Fernando Filoni (che anch'io ho contattato e con il quale sono stato in colloquio telefonico

per assumere l'incarico di sostituto alla Segreteria di Stato), si sono adoperate da allora per mantenere un costante flusso di informazioni nei due sensi, tenendo la famiglia di padre Bossi costantemente informata di tutti gli sviluppi. Sul piano diplomatico contiamo sulla fattiva collaborazione delle autorità filippine, cui abbiamo chiesto fin dal primo momento di adottare tutte le le possibili iniziative per la soluzione pacifica del caso, evitando azioni che possano compromettere l'incolumità dell'ostaggio. Questa dell'incolumità dell'ostaggio è la priorità in tutte le iniziative che il Governo sviluppa quando si trova di fronte a casi di sequestro di persona, come peraltro

se ricordo bene), in cui, tra l'altro, si evidenziava l'elemento dell'incolumità dell'ostaggio come priorità. Il Governo filippino ha confermato il suo massimo impegno, anche con il dispiego di un ingente numero di truppe impegnate nelle ricerche sul terreno, ed ha informato la nostra ambasciata sugli sviluppi del caso e sulle iniziative che vengono promosse sia a livello centrale, che a livello di autorità locale, per identificare i responsabili ed eventualmente conoscere le rivendicazioni per la liberazione di padre Bossi. La scorsa settimana il nostro ambasciatore a Manila si è recato a Zamboanga City per verificare direttamente la situazione con le autorità *in loco*, ricevendo conferma degli sforzi profusi nel promuovere ogni utile iniziativa per la liberazione del missionario. Su un piano più generale, ricordo che Mindanao è teatro da circa 500 anni di un conflitto tra la componente musulmana, presente sull'isola ben prima della colonizzazione spagnola, e la maggioranza cristiana, che fa riferimento al Governo di Manila. I musulmani sono attualmente una minoranza nella popolazione di Mindanao, e sono concentrati soprattutto in una regione autonoma che riunisce quattro province. Nonostante gli accordi di pace con il Governo, la situazione non ha ancora trovato nei fatti una composizione definitiva. L'opposizione musulmana è in prevalenza rappresentata dal *Moro National Liberation Front* fondato nei primi anni Settanta, con l'obiettivo di realizzare una patria musulmana a Mindanao. Alla fine degli anni Settanta, per problemi di *leadership*, si è separato dal *Moro Islamic Liberation Front* (MILF), che con circa 12.000 militanti riunisce l'*élite* intellettuale e della nobiltà tradizionale musulmana delle isole, i cosiddetti Datu, meno conciliante verso ipotesi di pace con il Governo e più attento alle tematiche religiose. L'estremismo islamico ha trovato una sua espressione locale nel movimento Abu Sayyaf, testualmente «colui che porta la spada», e che si ritiene collegato ad Al Qaeda e al movimento fondamentalista islamico indonesiano Jemaah Islamiya. I *moros* filippini (così sono denominati i musulmani di Mindanao dai tempi della dominazione spagnola) sono tradizionalmente temibili guerrieri. Alcuni di loro hanno militato in Al Qaeda fin dai tempi della guerra in Afghanistan negli anni Ottanta, ed hanno approfondito i legami con i vertici del jihaidismo internazionale, con periodi di comune formazione militare e religiosa in varie parti del mondo. Tali legami sono ancora oggi molto solidi. I gruppi sopra citati non sono tuttavia nettamente distinti. Numerosi sono i legami trasversali, familiari e di interesse che rendono la composizione dei vari movimenti molto fluida e porosa. Le *leadership* provengono tutte dallo stesso ceppo originario ed hanno familiarità l'una con l'altra. Sono anche presenti frange semidissidenti che si richiamano ai valori del MNLF e del MILF, organizzazione secessionista del Fronte Moro, ma che agiscono in realtà a scopo di lucro, come vere e proprie bande criminali, spesso sconfessate dalle *leadership* dei maggiori movimenti. Centinaia, va ricordato, sono ogni anno i rapimenti di ricchi uomini d'affari cinesi presenti a Mindanao. La situazione sul terreno, dalla descrizione che vi ho fatto, comprenderete che è alquanto complessa. Nonostante quanto riferito da alcuni organi di stampa, al momento non si conosce la matrice del sequestro, né sono pervenute alle autorità filippine, al PIME o all'Italia rivendicazioni o richieste di riscatto. Sono comunque attentamente vagliate e verificate tutte le informazioni che pervengono da diverse fonti. Continuiamo quindi a non potere escludere nessuna pista, né la matrice criminale estorsiva, né quella fondamentalista qaedista, che potrebbe essere ricondotta al gruppo estremista Abu Sayyaf, né la possibilità di un passaggio di mano dell'ostaggio tra i gruppi attivi nell'isola. Con la discrezione e la riservatezza necessaria a non compromettere gli sforzi attualmente in corso, il Governo continua con determinazione a lavorare in stretto coordinamento con il PIME e le autorità filippine per la liberazione di padre Bossi. un atteggiamento doveroso, analogo a quello che il Governo ha tenuto, tiene e terrà in ogni caso analogo, senza fare distinzioni tra persone, ruoli e luoghi e sempre privilegiando l'obbiettivo prioritario, che è quello di salvare una vita umana. Come richiesto anche dagli stessi familiari del missionario che più volte hanno richiamato tutti al senso di responsabilità e ad evitare polemiche, si è cercato di evitare ogni pubblicizzazione delle intense attività diplomatiche e di quelle degli altri attori istituzionali presenti sul campo, che anche in queste ore continuano il loro lavoro insieme alle autorità filippine. Anche ieri il vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri D'Alema ha presieduto alla Farnesina un'ulteriore riunione operativa, cui hanno preso parte tra gli altri il superiore del PIME, padre Zanchi, e il segretario generale del PIME, padre Mariani, per fare il punto sulla vicenda e concordare ulteriori iniziative. Il Governo ha inoltre accolto con apprezzamento, in ragione dei consolidati rapporti (che in qualche caso sono anche rapporti di amicizia personale, personale, maturati negli anni passati) la disponibilità dell'onorevole Boniver a recarsi nelle Filippine per contatti con le autorità locali. La missione dell'onorevole Boniver, accompagnata da funzionari dell'unità di crisi e dell'ambasciata a Manila, è attualmente in corso e auspichiamo che nell'ambito delle iniziative promosse dal Governo

Signor Presidente, ho chiesto di parlare solo per esprimere apprezzamento e solidarietà per quello che il Vice ministro ci ha detto e per quello che il Governo sta facendo. Occorre richiamare l'attenzione

prendessimo l'occasione di sottolineare un fatto a cui si presta pochissima attenzione e di cui non si parla mai.

una soluzione: Nasser dovette derogare dal fatto di volere per forza un arabo e si trovò un salesiano libanese che andasse a dirigere la scuola, e così la questione fu risolta. Mi pareva giusto dire una parola non solo nei confronti di questo missionario, ma per le missioni in genere. Signor Presidente, purtroppo non posso condividere l'apprezzamento del senatore Andreotti nei confronti del Governo, perché da quello che ci ha detto il vice ministro e senatore Danieli, che ringrazio per essere venuto in quest'Aula molto tempestivamente, la sensazione che avevamo nei giorni scorsi, cioè che ci fossero due pesi e due misure in funzione dei rapiti, ahimè, è purtroppo confermata. Oggi il Governo ci ha comunicato che non sappiamo nemmeno, e abbiamo vaghe idee, di chi abbia in mano in questo momento e di chi abbia rapito padre Bossi. A quasi un mese dal rapimento, questo mi pare un grave *deficit* di informazione e credo che la collaborazione con le autorità locali difetti quantomeno di conoscenze e di *intelligence* sul territorio. È ovvio e naturale che, trovandoci in uno Stato sovrano che non si trova in questo momento in una condizione di guerra, forse è difficile schierare i nostri uomini dell'*intelligence*, ma è altrettanto ovvio che quando il sistema politico, e anche parte del sistema istituzionale, massacra i nostri Servizi segreti, che bene hanno agito sul campo, è difficile che questi possano avere la credibilità e l'autorevolezza per poter lavorare. Ma c'è di più, signor Presidente, colleghi, signor Vice ministro,

al caso della giornalista Sgrena e ad altri casi - si è mobilitato non solo un Governo, non solo un Parlamento, ma un Paese, attraverso una grande forma di pressione popolare dei mezzi radiotelevisivi di massa, il sequestro di padre Bossi è stato letteralmente nascosto, ed è stata sequestrata anche la verità su di lui. Ieri si è tenuta una manifestazione popolare, promossa da un grande intellettuale di questo Paese,

silenzio ed anche il fatto che si è fatto un affare di Stato, dando priorità assoluta alla liberazione di un amico dei talebani, che era stato coinvolto nella liberazione del giornalista Mastrogiacomo, e non si dà lo stesso rilievo a un missionario, il quale ha forse il torto di non scrivere su "la Repubblica" o su "il manifesto". È vergognoso il fatto che tale manifestazione sia stata letteralmente censurata dal servizio pubblico televisivo e dal TG1, per la semplice ragione che vi erano presenti più esponenti dell'opposizione che dell'attuale maggioranza, ai quali non era preclusa la partecipazione, anzi era stata sollecitata. Una presenza un po' più massiccia degli esponenti della maggioranza avrebbe forse fatto in modo che anche il direttore del TG1 e delle altre testate che fanno riferimento alla maggioranza di Governo si rendessero conto dello scempio di verità, di conoscenza e di allarme nei confronti del popolo italiano che stanno compiendo. Ora, signor Vice ministro, lei ci ha esposto un'informativa puntuale per quanto le era possibile, ma devo dire - e mi rendo conto delle difficoltà a dare ulteriori notizie per non compromettere eventuali azioni in corso apprezzo anche il fatto che il Governo abbia gradito l'intervento di un esponente del Governo precedente. Mi chiedo però se non vi rendiate conto che avete bisogno di questo tipo di supporto, perché forse non siete in grado, o non avete la volontà, di impegnare tutte le forze che il Paese può mobilitare per liberare padre Bossi. Quando a Palazzo

devo dire che, al contrario del senatore Stracquadanio, apprezzo, come ha fatto il senatore Andreotti, le informazioni che ci ha comunicato il vice ministro Danieli. Lo dico con molta chiarezza e nettezza, perché non vedo né nelle

Per quanto mi riguarda, Giancarlo Bossi è uguale a Giuliana Sgrena ed avendo potuto conoscere tanti missionari che hanno lavorato e che lavorano, li sento non soltanto profondamente vicini a me ma anche a tutto il nostro popolo.

dalla dichiarazione del vice ministro Danieli, ma anche leggendo le notizie di tutti i giorni emerge cosa c'è a Mindanao: in quella situazione l'incolumità diventa il punto essenziale. Vogliamo farlo uscire vivo, io penso, e questo è decisivo: trovarlo vivo.

ma chiedo a tutti voi: servono le polemiche strumentali, che io leggo in modo strumentale? Non credo servano, perché l'obiettivo di tutti noi è quello di salvare una vita umana. Vorrei anche ricordare che, nei dibattiti che abbiamo avuto, in particolare quello dopo la liberazione del giornalista Mastrogiacomo, in quest'Aula fu proposto un ordine del giorno in cui non si metteva più al primo posto

ma non azioni che possano creare qualche problema. E' evidente anche che ci troviamo in una situazione complessa, dove forse è anche più difficile avere

di preghiera e anche altre iniziative per far conoscere il lavoro dei missionari, ma evitiamo strumentalizzazioni, perché l'obiettivo di tutti noi è riportare nella sua casa, ai suoi affetti e alla sua missione religiosa padre Giancarlo Bossi.

c'è oggi una persecuzione dei cristiani, di cui forse facciamo fatica a renderci conto. Dieci milioni di cristiani costretti ad emigrare dal Medio Oriente, dai Paesi islamici;

con chi in qualche modo fa discriminazione e uccide i cristiani; non possiamo continuare ad appoggiare il macellaio dell'Iran che mette sotto scacco Israele e minaccia tutto l'Occidente. Dobbiamo smetterla con questo buonismo, cominciando a difendere veramente quelli che stanno soffrendo in questo momento, smetterla di pensare di avere noi tutte le colpe dei mali del mondo e guardare in faccia a quanto sta accadendo. Chi sta tagliando le teste non è un gruppo piccolo non è un gruppo piccolo che fa parte del terrorismo, ma di una determinata mentalità verso cui noi siamo purtroppo accondiscendenti. Veniamo ora al Governo.

che urla al telefono: "Libere. Per i Torretta è la fine dell'incubo". Per Hanefi si usa il grimaldello di D'Alema. D'Alema interviene personalmente minacciando il Governo di annullare la Conferenza di Roma a Potsdam. Abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare? In passato, si è mosso Frattini, questa volta l'ex ministro Boniver che ringraziamo. Si può sinceramente dire che si è fatto tutto quanto era nelle nostre possibilità? Non lo so. Io non posso scagliare la prima pietra, però mi sembra di capire che il clima del Paese, l'entusiasmo, i livelli di Governo attivati in passato per le due Simone, per la Sgrena mancano; i Servizi segreti, purtroppo come diceva il collega Stracquadanio - non ci sono più o se ci sono non si fanno vedere, la Croce Rossa non c'è, la catena di comando si è sfilacciata. Su questo, signor Sottosegretario, credo che una qualche responsabilità o omissione, se non altro di entusiasmo e di partecipazione, questo Governo, ma anche gran parte del Paese ce l'abbia verso questo nostro fratello.

precisa. Non è mancato neanche un breve *excursus* sulla storia dei movimenti terroristici nelle Filippine, ma alla fine della relazione c'era qualcosa che non mi tornava. Mi sono detto: "Cosa c'è che non funziona?" Signor Vice ministro, mancava l'indignazione, mancava il sangue, mancava l'emozione, mancava la passione, mancava un giudizio politico. Questa non è un'assemblea di funzionari ai quali raccontare burocraticamente quello che il Governo sta facendo, ma un'assemblea politica che rappresenta la Nazione, la quale vuole un giudizio politico da parte del Governo. Mi scusi, ma io questo giudizio non l'ho ascoltato. Mi veniva in mente un passaggio dell'Amleto

Il senatore Andreotti ha dato un suggerimento su come si poteva impostare un giudizio politico, magari cominciando con il ricordare la grande opera di bene che i missionari italiani fanno in tutto il mondo, magari lanciando un messaggio ai rapitori per dire loro che questo è un uomo di pace, un uomo di bene, bene, un amico del popolo filippino, un amico degli ultimi, dei poveri, che non merita certo né la morte né la prigionia. Non l'ho sentito. Sarebbe stato utile, importante un appello del Governo italiano che ricordi la figura morale di padre Bossi ed esprima indignazione per

magari prendendo un impegno a nome del Governo sull'opportunità di mettere la difesa della libertà religiosa al centro della propria azione di politica estera. Che non capiti più che un Ministro italiano vada all'estero, in Paesi nei quali la gente soffre per la libertà religiosa o per altre libertà, per per trattare affari senza rivendicare il diritto alla libertà. Non chiedo mica la sospensione dei rapporti commerciali! Il Il presidente Andreotti ha omesso questo passaggio, ma è stato un maestro di questa politica. Si può, ogni volta che si va, agire concretamente. Non ho sentito nemmeno questo. Ci sono altri percorsi possibili. Si poteva inquadrare quanto è accaduto all'interno della guerra contro il terrorismo, affermando la determinazione dell'Italia di proseguire in questa guerra con un ammonimento: non toccate i cittadini italiani, perché chi toccherà cittadini italiani verrà sicuramente, inflessibilmente, perseguito, scovato, trovato e punito. Non ho sentito nemmeno questo. Mi domando, allora, qual è il giudizio politico del Governo su quanto accaduto e quali sono gli impegni politici che il Governo prende davanti a noi: l'impegno di dire al rappresentante diplomatico *in loco*, all'unità di crisi di fare tutto il possibile? Questo sicuramente lo faranno. Ho grande fiducia nel senso del dovere e anche nelle capacità dei nostri funzionari;

come sindaco di Roma prima ancora che come prossimo Presidente del Consiglio per conto della coalizione di maggioranza. Non ho visto Ministri del Governo a quella manifestazione e forse sarebbe stato bene che fossero stati presenti. Non ho sentito, signor Vice ministro - non è una critica personale a lei, ma una critica politica a questo Governo - la determinazione, la passione, la capacità di esprimere un giudizio politico, la volontà decisa, non genericamente di fare tutto il possibile,

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, chi ci guadagna dal rapimento di un prete? Cosa può aver spinto a privare della libertà padre Giancarlo Bossi, un uomo la cui generosità è pari alla sua mole fisica? È un rapimento a sfondo ultrafondamentalista? È un prete, fa del bene al prossimo, non partecipa ad attività politica. È un rapimento a scopo di estorsione? E' un prete, non ha soldi, né lui, né la sua famiglia, né il PIME; anzi, normalmente si raccoglie denaro per mantenere le missioni, soprattutto in quelle zone a rischio sconsigliate dalla Farnesina. Non si capisce il perché e non si capisce il come. Finora non ci sono prove neanche che padre Bossi sia in vita. Condivido l'appello dei familiari di padre Giancarlo e del PIME a non creare ostacoli, neanche involontariamente, per il suo rilascio con polemiche e con divisioni politiche. Oggi è il momento dell'unità politica ed istituzionale, tesa a liberare un nostro connazionale che è in pericolo. Anch'io ringrazio il rappresentante del Governo per l'informativa e spero, anzi sono convinto, che le sue parole non fissino graduatorie di durata dei rapimenti: che altri siano durati sei mesi o tre mesi è assolutamente irrilevante. Leggo da una agenzia Reuters di oggi che l'esercito delle Filippine sta cercando padre Bossi con duemila uomini - così dice il generale Esperon dell'esercito filippino Esperon dell'esercito filippino - e che alle ricerche si sono aggiunte alcune dozzine di militari addestrati dagli Stati Uniti d'America. Mi chiedo perché non si ha notizia di uomini dei nostri Servizi, che forse potrebbero dare un utile contributo informativo, e non solo, se qualcuno li lascia operare in pace. Ciò che è indispensabile è che il Governo italiano prema costantemente sul Governo filippino perché sia chiaro che il rapimento di padre Bossi - come prima ricordava il presidente Buttiglione - non è una pratica diplomatica, ma qualcosa a cui il popolo italiano tiene in modo particolare. Forse, affinché ciò sia ancora più chiaro, potrebbe essere utile un'informativa periodica (scegliete voi, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, il grado di periodicità: settimanale, ad esempio, e speriamo non sia necessaria una periodicità superiore) al Senato, magari in un orario che consenta una partecipazione più ampia dei colleghi. Insieme a ciò - mi riallaccio alle parole dei colleghi che sono intervenuti prima l'istituzione, in seno al Governo, di un comitato che monitorizzi in permanenza la situazione della libertà religiosa nel mondo, che è il fondamento di tutte le altre libertà. Ieri sera - lo si ricordava prima - l'immagine di padre Bossi campeggiava nella piazza Santi Apostoli nella manifestazione "Salviamo i cristiani", a sollecitare pubblicamente la sua liberazione. Sono certo che più se ne parla, più si preme sulle autorità filippine e più è possibile che si attivino tutti i canali per giungere all'esito sperato. sperato. Signor Presidente, non so chi guadagna dal rapimento di un prete; so, però, che cosa si perde se non sarà liberato. Ciascuno di noi perderà se il sequestro non si concluderà positivamente, qualunque sia la confessione religiosa di appartenenza e anche se non apparteniamo a nessuna confessione religiosa. Tutti dobbiamo sentirci impegnati, Governo in testa, in questa direzione, anche a vincere l'indifferenza e il silenzio. Ho riletto con un brivido i versi del pastore protestante Martin Niemöller, morto a Dachau. «Prima vennero per gli ebrei, e io non dissi nulla perché non ero ebreo. Poi vennero per i comunisti, e non io dissi nulla perché non ero comunista. Poi vennero per i sindacalisti, e io non dissi nulla perché non ero sindacalista. Poi vennero a prendere me e non era rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa». signor Presidente, in tutto il mondo vengono per cristiani, sacerdoti, religiosi e laici, ma se non c'è nessuno che dice qualcosa, poi verrà l'ora degli altri. È solo un problema di tempo. Per questo l'ora di padre Bossi va sentita come l'ora di tutti. *(Applausi

celerità su questa vicenda e voglio garantire da parte di Forza Italia tutto l'appoggio per l'attività che certamente il Governo sta svolgendo per arrivare alla liberazione di padre Giancarlo Bossi, come è testimoniato dalla presenza sul posto della nostra collega, l'onorevole Margherita Boniver. Detto questo, credo vadano svolte alcune considerazioni politiche di carattere generale. Indubbiamente, infatti, la situazione che si è venuta a creare

dal Governo afghano alcuni terroristi per ottenere la liberazione del giornalista Mastrogiacomo, non sia stata la giusta via per scoraggiare e per prevenire altri terroristi dal rapire altri cittadini italiani. Far mancare l'appoggio agli uomini del SISMI, com'è avvenuto in questi mesi, non è la via giusta per incoraggiare quegli uomini - che lavorano sul campo,

sia di carattere giuridico. Far marcare loro ogni appoggio, lasciandoli in balia di inchieste che francamente lasciano perplessi, non è un buon modo per scoraggiare coloro che possono scoraggiare coloro che possono pensare di rapire un cittadino italiano, o più in generale qualunque cittadino inerme, perché naturalmente non dobbiamo pensare solo ai cittadini italiani; non è un buon modo per avere i nostri uomini pronti, operativi ed efficaci nel momento in cui dobbiamo chiedere loro di rischiare la vita. Ricordo che il ruolo dei Servizi segreti è stato fondamentale nella liberazione di altri ostaggi e il sacrificio di Nicola Calipari, uomo dei Servizi, per

riflettevo sul fatto che è incredibile che occorra una manifestazione, promossa da un coraggioso giornalista, peraltro di religione musulmana,

far sentire la sua positiva vicinanza agli uomini che rischiano in circostanze simili; credo sia compito del Governo far sapere - come è stato detto molto bene dai colleghi che sono intervenuti prima di me - che non

per i gruppi terroristici delle Filippine, ma soprattutto - e può valere più facilmente, perché sono di certo più facili da individuare come referenti - vale nei confronti dei Governi di quei Paesi

Signor Presidente, ringrazio il vice ministro Danieli per le informazioni che ci ha dato e lo ringrazio anche per il per il riserbo con cui ha trattato i particolari della questione su cui stiamo discutendo oggi in Senato. Credo che i sequestri di persona, soprattutto quelli di questo tipo, vadano trattati, finché non sono terminati, con grande prudenza. Ringrazio il Governo di averlo fatto e sono certo che il Governo tornerà in Senato quando, come noi ci auguriamo, il sequestro sarà concluso con la liberazione di padre Bossi e, in quelle circostanze, conosceremo anche tutti i particolari dell'azione che i nostri Servizi di sicurezza, i nostri Servizi segreti il nostro corpo diplomatico hanno svolto per liberare padre Bossi. Ho sentito anche rassicurazioni sul fatto che non esistono, per il Governo italiano, sequestri di prima e di seconda categoria. Non avevo bisogno di sentirlo, ero certo che così fosse, credo che questa sia una convinzione unanime del Parlamento. So, come tutti noi sappiamo, che esiste in realtà il pericolo che i sequestri vengano diversamente valutati a seconda delle Regioni dove avvengono e che sia possibile, effettivamente - ma questo è un problema che riguarda la cultura dei *media* e una certa cattiva politica - che i sequestri che avvengono in Iraq piuttosto che in Afghanistan vengano considerati più importanti di quelli che avvengono nelle Filippine. Credo che questo sia sbagliato; so che il nostro Governo non cade in questo errore. Purtroppo sono caduti in questo errore alcuni *media* e francamente me ne dispiace, soprattutto dove ho letto, in questa disparità di trattamento, di approfondimento e di valutazione, uno spirito politico negativo che, in queste circostanze, dovrebbe essere sempre assente. Vorrei svolgere, però, due considerazioni di carattere generale che hanno espresso in parte già i colleghi. La prima: io vorrei ricordare al Senato che negli ultimi due decenni la sicurezza nel mondo è molto cambiata. Oggi sono in atto, mentre noi parliamo, centinaia di piccole e medie guerre, piccole e medie rivolte, tensioni, scontri, ogni volta con gravi rischi anche di sequestri di persona. uno sviluppo tragico e, dal mio punto di vista, terribile di grande criminalità internazionale, anche questa condita con sequestri di persona, forme di schiavitù, traffico di organi umani. Credo che sia un imperativo per tutti i Governi, e so che lo è anche per il nostro, cercare di ridare stabilità e un ordine internazionale. L'unica maniera in cui possiamo sperare di frenare questo fenomeno è proprio cercare un nuovo equilibrio internazionale, un nuovo modo di relazionarsi tra gli Stati. ripensare veramente all'organizzazione delle Nazioni Unite, all'Unione Europea, cercando di dare a questi grandi organismi non soltanto l'autorevolezza, ma anche la forza che serve per intervenire in questi fenomeni che stanno modificando e straziando il nostro pianeta. La seconda considerazione è stata svolta già prima dal presidente Andreotti e poi anche dai colleghi che sono intervenuti, il senatore Polledri, il senatore Mantovano e, da ultimo, anche dal senatore Malan e riguarda il ruolo della Chiesa e il ruolo delle missioni. Noi oggi abbiamo una grande ammirazione e gratitudine per le ONG, per le organizzazioni di gratitudine per le ONG, per le organizzazioni di volontariato, ma la Chiesa, con le sue missioni, è stata forse la prima grande forma di globalizzazione umanitaria del mondo.

celebrò, per la prima volta nella storia della Chiesa, i nuovi martiri, ricordando al mondo che i martiri cattolici del '900 hanno hanno superato per numero - lo ha ricordato anche il senatore Polledri - addirittura i martiri dei primi secoli della Chiesa cattolica. Ma il Papa non ha parlato, citando i martiri del '900, di martiri provenienti dalla lotta tra l'Islam ed il cattolicesimo. Non ha parlato di questo, perché non è questo lo spirito del martirio della Chiesa, che è piuttosto nello spirito di missione che ispira le missioni della Chiesa cattolica. Mi piace ricordare le parole con cui Papa Wojtyla ha parlato dello spirito delle missioni, quando ha ricordato - durante il Giubileo del 2000 - come l'atteggiamento missionario inizia sempre con un sentimento di profonda stima di fronte a ciò che c'è in ogni uomo e che la Chiesa è sempre solidale con le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. Ed è per questi motivi, per questo modo di intendere la missione dei dei preti e dei missionari, che io credo che il rapimento di padre Bossi umili veramente in modo particolare chi l'ha commesso.